per inquadrare e chiarire la questione, per la verità un po' complessa, conviene ripercorrere brevemente la storia della scuola IMT Alti studi di Lucca. Nell'ambito della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 il Ministero stipulò un accordo di programma con il Consorzio interuniversitario di studi avanzati, detto CISA, costituito dal Politecnico di Milano, dalla Scuola Sant'Anna di Pisa e dalla Libera Università LUISS di Roma, per la realizzazione di una scuola di dottorato di ricerca, denominata IMT, con sede a Lucca, con il requisito di una partecipazione significativa di istituzioni lucchesi. Un gruppo di istituzioni lucchesi (Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Fondazione banca del monte di Lucca, Associazione degli industriali della Provincia di Lucca e

con l'Università di Pisa, ateneo di riferimento del territorio, per la realizzazione della nuova scuola di dottorato IMT. Tale scuola cominciò a funzionare nel marzo 2005 potendo contare, da un lato, sui finanziamenti ministeriali del piano triennale 2004-2006 assegnati al Consorzio CISA in base all'accordo di programma e, dall'altro, sui finanziamenti e sulle strutture logistiche messi a disposizione dalla citata Fondazione. Con decreto ministeriale del 18 novembre 2005 la Scuola IMT viene istituzionalizzata. In altri termini, viene istituita la scuola IMT Alti studi di Lucca come istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale sulla base di uno statuto contenuto nel medesimo decreto. Il mese successivo, con l'approvazione del maxiemendamento alla legge finanziaria per il 2006, venne assegnato alla nuova istituzione universitaria un contributo ordinario di funzionamento pari a 1,5 milioni di euro. Su tali atti governativi si aprì subito una vivace polemica politica, centrata sulla repentina costituzione ufficiale di una università di eccellenza proveniente da una scuola di dottorato che aveva meno di un anno di vita. All'acceso dibattito, che si protrasse per tutta la campagna elettorale per le elezioni politiche del 2006 e oltre, partecipò, tra gli altri, il professor Luciano Modica, allora senatore della Repubblica e poi candidato alle elezioni del Senato per il collegio della Toscana.

di Pisa per l'annullamento del decreto ministeriale di costituzione della scuola IMT Alti studi di Lucca, riscontrando a suo giudizio il mancato rispetto di alcune clausole delle convenzioni stipulate che prevedevano una partecipazione della Fondazione agli organi di governo della scuola. A questo punto, di fronte al ricorso della fondazione FLAFR, la Scuola IMT entra in una fase di stallo e tutte le attività vengono bloccate dal Consiglio Provvisorio dell'IMT. Il medesimo Consiglio chiede al direttore del consorzio CISA, professor Gaetano Quagliariello, di trovare un nuovo accordo con la Fondazione, ma il testo di nuovo statuto, preparato, tra l'altro, con la mediazione del professor Giulio Ballio, rettore del Politecnico di Milano (uno degli atenei aderenti al CISA), non trova il consenso del direttore del CISA, che propone altri emendamenti (i quali, di fatto, snaturano i termini essenziali dell'accordo e con cui, comunque, si impedisce, a questo punto, agli enti aderenti alla FLAFR di convergere su di una soluzione collaborativa tale da consentire il ritiro del ricorso). nonostante, il 23 febbraio 2006, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del tempo stipula con la Scuola IMT un accordo di programma che prevede un contributo finanziario a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università, in aggiunta a quello già stabilito dalla legge finanziaria 2006, «in correlazione con l'andamento del fondo per il finanziamento ordinario e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 56, comma 5, della Questa è la situazione di fronte alla quale si è trovato il nuovo Ministro dell'università e della ricerca, insediatosi dopo le elezioni politiche del maggio 2006. Questi, con l'obiettivo di facilitare la soluzione dell'*impasse* istituzionale venutasi a determinare con il ricorso della Fondazione e di porre i presupposti per il pieno sviluppo della scuola IMT, risolvendo il conflitto creatosi tra le istituzioni fondatrici, incarica il neosottosegretario Modica di aprire e coordinare un tavolo di mediazione fra tutti gli attori della vicenda. L'obiettivo è assicurare il raggiungimento di un accordo che definisca un profilo accademico chiaro e stabile alla nuova autonoma istituzione universitaria di eccellenza nell'ambito del sistema universitario toscano e nazionale; di caratterizzare in modo innovativo e sperimentale (soprattutto dal punto di vista della *governance* e della docenza) la Scuola IMT; di recepire il notevole e positivo impegno messo in campo dalle istituzioni del territorio di Lucca; di garantirne lo sviluppo in base alle risorse assegnate dalla legge e fornite dalla Fondazione. Peraltro, nel territorio della Toscana nordoccidentale - com'è noto - opera già il sistema universitario pisano, formato dall'Università di Pisa e dalle due storiche Scuole universitarie di eccellenza costituite dalla Scuola Normale Superiore e dalla Scuola Sant'Anna. Il 7 agosto 2006, il Ministro, con una nota indirizzata al presidente della Scuola IMT, comunica che, «non essendo al momento noto quale sarà l'andamento del fondo di finanziamento ordinario per i prossimi esercizi in relazione alle esigenze complessive del sistema universitario, si invita la Scuola a non prendere in considerazione, nel proprio bilancio di previsione 2007, importi relativi all'attuazione di tale accordo», ovverosia dell'accordo di programma del 23 febbraio 2006, e fa inoltre presente che «i contenuti del predetto accordo saranno oggetto di ulteriori approfondimenti anche ai fini di una rinegoziazione dello stesso». Il tavolo di lavoro intanto coordinato dal sottosegretario Modica, riunitosi nei mesi di luglio e settembre, giunge, nell'ottobre 2006, con l'adesione unanime di tutti i partecipanti, a stendere una bozza di nuovo statuto della Scuola IMT. Recepiti tutti i pareri di rito delle istituzioni universitarie e territoriali coinvolte, il 23 novembre 2006 il nuovo statuto della Scuola IMT è stato approvato all'unanimità dal Consiglio provvisorio della scuola Sulla base della deliberazione assunta, lo statuto è stato successivamente emanato dal direttore della scuola, in data 6 febbraio 2007, e pubblicato sulla *Gazzetta* *Ufficiale* del 22 febbraio. Il nuovo statuto è entrato in vigore il 9 marzo scorso; immediatamente, la fondazione FLAFR ha attivato il ritiro del ricorso al TAR. Con l'insediamento del nuovo Consiglio direttivo, in corso di completamento, e con la nomina, da parte dello stesso, del nuovo direttore, l'attività della Scuola IMT potrà riprendere a pieno ritmo, anche se occorre riconoscere che, per il contributo continuo della fondazione FLAFR, del direttore uscente, dei coordinatori dei corsi e degli uffici della Scuola, l'attività didattica, amministrativa e gestionale, comunque, è proseguita correttamente, anche durante il periodo di crisi istituzionale. Venendo ora ai quesiti specifici degli onorevoli interroganti, il Ministro della ricerca risponde che, con il nuovo Statuto, è stata ristabilita - in piena legalità e con il consenso unanime delle università e delle istituzioni impegnate nel progetto - la completa funzionalità della Scuola IMT e che, di conseguenza, la Fondazione ha ritirato il ricorso presentato al TAR della Toscana. Per quanto riguarda il rispetto del principio dell'autonomia didattica e dell'autonomia universitaria in generale, si desidera rassicurare i senatori interroganti sul totale rispetto di questi principi, in quanto, peraltro, il nuovo statuto della Scuola IMT, all'articolo 1, comma 1, afferma che la Scuola IMT è «un istituto statale di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale» - quindi come era - «inserito nel sistema universitario italiano, dotato di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile». Il nuovo statuto prevede un impianto di *governance* incentrato attorno a un consiglio direttivo e a un collegio accademico. Il consiglio direttivo è composto da sei rappresentanti designati dalle università

composizione del Consiglio direttivo non preveda alcun particolare ruolo delle istituzioni universitarie pisane, da un altro come la Scuola consideri quali *partner* naturali la Fondazione FLAFR. Il ritiro del ricorso al TAR, d'altra parte, mostra la piena soddisfazione della Fondazione che rappresenta gli interessi della città di Lucca. Per completezza di informazione occorre aggiungere che, con nota aggiuntiva allo Statuto, sono già previste le modifiche da apportarvi nel caso in cui la Scuola Normale Superiore accogliesse l'invito ad aderire al progetto scientifico ed organizzativo della Scuola IMT. Per quanto riguarda, infine, la questione dell'accordo di programma firmato il 23 febbraio 2006, è stata già indicata l'azione del Ministro per ricondurlo alla corretta applicazione delle norme riguardanti l'utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario delle università statali per il 2007 una volta che l'entità definitiva e le condizioni di contesto del sistema universitario siano note. Infatti il decreto di ripartizione del fondo

Nella mia interrogazione avevo chiesto se il Ministro non ritenesse opportuno smentire le dichiarazioni dell'attuale sottosegretario per l'università, Luciano Modica. lei ha parlato della campagna elettorale alla quale ha partecipato lo stesso Modica. Posso capire che in campagna elettorale qualche dichiarazione dettata dalla passione politica scappi di mano, anzi, nella fattispecie, di voce. Ma alcune dichiarazioni sono state rilasciate dopo la campagna elettorale. Cito «Report»: secondo Modica, l'IMT era un regalo elettorale a potentati locali. Cito «l'Unità di Firenze» della Toscana

di un disegno teso a denigrare l'IMT, in accordo con altri istituti della Regione ed evidentemente anche in accordo con gli enti locali, che non vedevano l'ora di poter insediare qualche loro rappresentante all'interno della Scuola. Non sono soddisfatto, signor Sottosegretario, anche perché nella mia interrogazione avevo chiesto se il Ministro intendesse ristabilire una situazione di normalità e di legalità. Non si può riconoscere formalmente l'IMT come istituzione universitaria autonoma e non tutelarne poi l'autonomia didattica e, anzi, darle addosso come ha fatto il Non si può riconoscere l'IMT come istituzione universitaria autonoma e poi agire fuori della legge. I docenti dell'IMT non sono più tali, sono in realtà tutti distaccati. La composizione del Consiglio di amministrazione dell'IMT vede una presenza paritaria delle rappresentanze locali.

Berlusconi aveva finanziato l'IMT; il Governo Prodi, con la sua finanziaria, ha tolto ogni risorsa all'IMT. Oggi la verità è che, finito il Governo Berlusconi, è finito il bel sogno di fare dell'IMT un centro di eccellenza nel mondo della ricerca e nel campo della formazione dottorale. Oggi l'IMT è ridotto a una modesta cosa locale, in mano a clientele politiche,

circa da quando sono state presentate le interrogazioni, avrei preferito che a rispondere fosse un Sottosegretario del Ministero competente. Non è la prima volta - credo non sia neanche l'ultima - che si ricevono degli atti di scortesia anche dal punto di vista istituzionale.

Quando l'IMT nacque, il primo bando ebbe oltre 1.000 domande, gran parte delle quali provenienti dall'estero. Era uno dei pochi casi in Italia nel quale si realizzava un percorso inverso: all'IMT si importavano cervelli e non si esportavano. Iniziarono subito i tentativi di far fuori questa piccola particolarità nel mondo accademico che evidentemente non rispondeva né a dei criteri accademici, né ai criteri politici preminenti all'interno della Regione. E questo non perché l'IMT fosse una scuola di diverso orientamento ideologico.

Ichino, Vittorio Strada, Aldo Schiavone, Sabbatucci e Zingales. Non mi sembra siano nomi che si possano riferire ad uno schieramento politico,

di Firenze, un esponente della Margherita. Cosa accadde a quel punto di fronte a questo inatteso successo? Nel momento in cui fallì il tentativo di far chiudere la scuola con un attacco diretto, si cercò di conquistarla casamatta dopo casamatta. Il disegno è descritto perfettamente nel documento che la Scuola Sant'Anna inviò al Ministero, in cui è detto in quale modo si sarebbe dovuta "normalizzare" l'IMT, alcuni stralci del quale sono stati riportati nell'interrogazione. Mi permetta di sintetizzare perché il tempo non mi consente di essere più specifico: si trattava appunto di ridurre la scuola ad una *dépendance* del polo pisano, negandole ogni originalità scientifica e negandole quel meccanismo di sedimentazione del sapere, che è garanzia di autonomia ed insieme di autorevolezza. Per chiunque lavori nell'università questo è pane quotidiano. Nel corso della campagna elettorale - lo ha detto lei - l'odierno sottosegretario Modica si distinse per aver partecipato a questa campagna, affermando cose che, con un eufemismo, possono essere definite delle inesattezze e che come tali sono documentabili.

nel documento, i cui stralci sono riportati nell'interrogazione. Lei dice che non c'è da temere per il rapporto di tipo particolare con le università pisane. Lei si immagina che nello statuto di una scuola superiore di Oxford vi sia un articolo che disciplini il modo nel quale quella scuola si deve

In linguaggio storico questo si chiama colonialismo di fatto, che è solo un po' differente da quello che si applica in maniera palese e quantomeno più onesta. Vi è ancora di più perché questo statuto nega la possibilità che vi siano docenti di ruolo in questa scuola. In questo modo si vìola una precisa previsione di legge: ciò che è stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Lo statuto, sotto questo aspetto, è illegale.

consiglio direttivo provvisorio, non ha consentito, non per una ragione di carattere ideologico, ma perché ciò non è permesso dalla legge. È contro la legge. Sotto questo aspetto si va ancora più in là e si fa qualcosa di ancora più grave, perché l'articolo 7 prevede che in Cda vi siano sei rappresentanti della FLAFR, dell'istituzione lucchese, e sei rappresentanti delle università. Quindi, apparentemente, vi è un rapporto paritario.

L'arcano è specificato all'articolo 10, lettera *b)*, nel quale si afferma che la mancata designazione ed elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio. due membri accademici "aggregati" quel collegio funzionerà con sei rappresentanti dell'ente privato di Lucca e quattro solamente dell'ente pubblico, in palese violazione di legge. Siamo in presenza di una falsa pubblicizzazione, che viola la disposizione secondo la quale lo Stato può finanziare al massimo per il 33 per cento le università o gli istituti superiori che contravvengono a quanto previsto per le istituzioni di natura statale. Vorrei per curiosità sapere di tutto ciò cosa ne pensa Rifondazione Comunista, che è tanto attenta all'interno del vostro Governo ad

per le quali il distacco da ciò che è previsto per le istituzioni statali è pagato, e a caro costo, con il fatto che non possano ricevere dallo Stato più del 33 per cento dei contributi per il loro funzionamento. Sia chiaro, per noi non è un problema ideologico, è un problema di legalità. Questo statuto è palesemente contro la legge. Mi chiedo se i dirigenti del Ministero se ne sono accorti e se hanno o meno sottoscritto questo statuto. Lo chiarirò con un'apposita interrogazione. Due problemi finali. della Scuola sono stati bloccati per due anni e non sono più arrivati dottorandi dopo quel bando eccezionale del 2005? è avvenuto in quanto non si poteva riunire il consiglio provvisorio, ma lei oggi ci ha detto che il consiglio provvisorio si è riunito anche in mancanza del suo presidente,

Infine (come vede io le accuse le formulo ad alta voce), è giunta in tutta Lucca una lettera firmata Unione cittadina amici di Lucca,

Presidente, in relazione all'atto parlamentare in esame si ritiene anzitutto opportuno premettere che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n. 103, non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte concernente la programmazione televisiva. Come è noto, infatti, la menzionata legge ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'attività governativa per assegnarla alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi televisivi la quale determina gli indirizzi dei vari programmi, vigilando sul contenuto degli stessi ed adottando, qualora se ne manifesti la necessità, le deliberazioni ritenute necessarie ai fini dell'osservanza degli indirizzi medesimi. Ciò premesso il linea generale, per quanto concerne la puntata andata in onda il 28 maggio 2006, del programma «Report» la predetta società RAI - interessata al riguardo ha precisato che il servizio nel dare conto dell'inaugurazione dell'Istituto IMT di Lucca, avvenuta nel precedente mese di marzo, e del finanziamento pubblico di 1,5 milioni di euro l'anno di cui il suddetto istituto beneficia, ha evidenziato il fatto che a fronte a fronte del finanziamento di nuovi istituti di ricerca, venivano tagliati i fondi per la ricerca delle università pubbliche. Nell'occasione, ha sottolineato la RAI, l'ex rettore dell'università di Pisa, solo successivamente nominato alla carica di Sottosegretario al Ministero dell'università e ricerca, ha espresso liberamente la propria opinione, mentre l'allora ministro dell'istruzione Letizia Moratti non ha concesso alla redazione del programma «Report» l'intervista che le era stata richiesta in data 27 febbraio 2006. Relativamente alla circostanza che la trasmissione in parola è andata in onda il giorno 28 maggio 2006, giorno dedicato al silenzio della campagna elettorale in quanto precedente lo svolgimento della votazione nel comune di Milano, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) cui spetta, ai sensi della legge n. 249 del 1997, il compito di garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di propaganda elettorale, ha comunicato quanto segue. I fatti addebitati alla signora Moratti, candidata alla carica di sindaco del Comune di Milano, peraltro attinenti al precedente incarico di Governo come titolare del Dicastero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, ed in particolare ad un finanziamento concesso alla scuola di eccellenza IMT di Lucca, non sembrano riconducibili alla campagna elettorale amministrativa e, pertanto, non sono assoggettabili alle disposizioni poste a garanzia del corretto svolgimento dell'informazione politica. II caso rappresentato non sembra rientrare, secondo l'avviso espresso dall'AGCOM, in nessuna delle tre tipologie contemplate dalle disposizioni vigenti in materia di programma di informazione: presenza dei candidati nelle trasmissioni di informazione, trattazione delle questioni relative alla campagna elettorale senza la partecipazione diretta di candidati, programmi di approfondimento informativo nei quali assume rilievo l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche. In merito alla asserita lesività delle affermazioni effettuate nel corso della trasmissione la suddetta Autorità ha comunicato di ritenere che la questione rientri nell'ipotesi della rettifica televisiva disciplinata dagli articoli 4, comma 1, lett. *e)* e 32 del Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 2005) e non nell'assenza di contraddittorio, ciò in considerazione sia della denunciata non veridicità dei fatti esposti -secondo quanto asserito dall'interrogante - sia del carattere della trasmissione, definita «giornalismo di inchiesta». Le norme suddette prevedono che chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie alla verità richiedere la rettifica all'emittente che ha trasmesso tali notizie e, solo in caso di esito negativo, inoltrare la richiesta all'Autorità per l'avvio dell'istruttoria procedimentale. In proposito, l'Autorità ha comunicato di non aver ricevuto, a tutt'oggi, segnalazioni di intervento in merito ai fatti oggetto dell'atto ispettivo in esame, ai fini del successivo avvio della rettifica.

È al corrente di chi era l'altro rappresentante della LUISS, della università nella quale ero professore universitario, nel Consorzio? Era l'attuale sottosegretario Gobbo, suo collega, così come altri suoi colleghi erano professori all'interno di quell'università. È al corrente soprattutto che tutto ciò che fu fatto per l'IMT, per la Scuola di Lucca, dal ministro Moratti in collusione, secondo il professor Modica, con il presidente del Senato Pera, fu anche previsto per l'Istituto italiano di scienze umane di Firenze, così come ha attestato poco fa il sottosegretario D'Andrea? Sa chi era il presidente di quell'Istituto? Un tale professor Umberto Eco che voleva lasciare l'Italia perché era stata soggiogata da un Governo criptofascista o qualcosa del genere. Queste sono state le irregolarità che sono state compiute a proposito di IMT; questi sono stati gli atti di parzialità che sono stati denunziati in quel servizio! Quando è andato in onda il servizio c'era già il Governo Prodi e il sottoscritto, così come l'allora presidente Pera, erano semplici senatori, laddove invece chi ci accusava era membro autorevole di quel Governo. Si è invertito il rapporto tra i poteri; di solito è il Parlamento che controlla il Governo e non viceversa. Per ragioni di stile, non fosse che per ragioni di Costituzione, quella trasmissione andava quantomeno evitata o aggiornata. La data nella quale certe cose sono prodotte non ha alcun senso, vale quando vengono offerte in pasto ai telespettatori, a centinaia di migliaia di nostri cittadini. Questa è evidentemente la concezione che alcuni membri del Governo hanno del pluralismo nel servizio pubblico. Non ci stupiamo se la legge Gentiloni che avete preparato è un caso emblematico, e resterà alla storia, come un esempio di analfabetismo legislativo.

cercherò di ricostruire molto dettagliatamente le procedure che sono state adottate perché è su questo punto che si incentra fondamentalmente l'interrogazione del senatore Amato. In previsione dell'organizzazione dell'evento culturale e promozionale «Primavera italiana 2007» in Giappone, un evento al quale il Ministero dei beni culturali partecipa con molteplici presenze, fu trasmessa da parte dell'ambasciata italiana a Tokyo, anche questo viene ricordato dal senatore Amato, da parte dell'ambasciatore Bova, la richiesta di prestito temporaneo del dipinto «Annunciazione»,

La Direzione generale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico incaricò il soprintendente *pro tempore* al polo museale fiorentino di seguire l'*iter* progettuale e organizzativo della mostra. Direzione generale, d'intesa con la Soprintendenza al polo museale, incaricò poi il personale tecnico di recarsi a Tokyo per visionare gli ambienti individuati per ospitare la mostra al fine di verificarne gli *standard* di sicurezza, microclimatici ed ambientali. Il sopralluogo permise di constatare la idoneità totale della sede espositiva. A cura della Soprintendenza per il polo museale fiorentino fu predisposta una relazione tecnica in cui stata evidenziata la stabilità conservativa dell'opera che - adottate le opportune precauzioni - ne rende possibile lo spostamento: è una citazione dalla relazione tecnica che faccio. La stessa Soprintendenza ha valutato positivamente l'opportunità del prestito che, pur diminuendo l'offerta della Galleria degli Uffizi, avrebbe ampliato, in sede internazionale, la conoscenza e l'apprezzamento per l'arte italiana, con conseguenti effetti benefìci sul turismo d'arte e dunque espresse parere favorevole al prestito. Acquisito il parere favorevole della Soprintendenza, la Direzione generale trasmise la richiesta di prestito al Comitato tecnico scientifico per il patrimonio storico artistico ed etno-antroplogico per le valutazioni di merito. Il Comitato, preso atto del parere favorevole, ha dettato una serie di condizioni di carattere tecnico atte a salvaguardare la sicurezza e la conservazione dell'opera ed ha espresso l'indicazione che il prestito di opere di valore venga in futuro bilanciato da scambi in regime di reciprocità, cui lei, senatore Amato, fa riferimento. La competente Direzione generale ha autorizzato il prestito a condizione che venissero adottate tutte le misure atte alla corretta conservazione sia nel trasferimento che nella conservazione dell'opera, ivi compresa l'assicurazione «da chiodo a chiodo, comprensiva dei rischi derivanti da atti di guerra non dichiarata e da terrorismo», cito il passaggio tecnico. E' stato inoltre richiesto l'interessamento del Prefetto, affinché, in occasione dello spostamento sul suolo nazionale, mettesse in atto ogni accorgimento necessario, ivi compreso quello della secretazione. Analoga richiesta è stata avanzata dal Soprintendente al polo museale, che ha chiesto la scorta armata, poi concessa, da parte del nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, tant'è che, come tutti ormai sappiamo, l'opera è giunta a Tokyo in condizioni tecniche dimostratesi felici. Al fine di garantire la massima sicurezza dell'opera sono stati adottati i più avanzati accorgimenti tecnici per l'imballaggio e per l'esposizione nella sede museale giapponese: triplice cassa con sensori offerti da due laboratori, uno italiano ed uno giapponese; vetrina speciale climatizzata e blindata costruita dalla migliore ditta esistente nel campo in Europa, la Glasbau Hahn di Francoforte sul Meno; è stato inoltre predisposto uno schema di protezione da parte dell'Arma dei carabinieri.

trasportata nel 1940 alla Villa dì Poggio a Caiano, poi a Camaldoli il 31 ottobre dello stesso anno e tornata agli Uffizi il 17 giugno 1945, dove fu esposta a partire dal 24 giugno 1948.

è altrettanto vero che questa tipologia di scambi può non limitarsi in modo rigidamente paritetico al solo ambito di «opera/oggetto d'arte». In materia di tecnologia, risorse e *know how* il Giappone può infatti offrire moltissimo alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico artistico italiano. Sono già in corso, peraltro a Firenze, dei progetti con grandi compagnie nipponiche, Hitachi e Nikon, che stanno portando ad un avanzamento tecnologico in alcune metodologie chiave della conservazione e della diffusione dell'immagine. Si potranno dunque creare ulteriori condizioni favorevoli a forme di intervento e collaborazione da parte di enti privati e pubblici giapponesi, ecco la reciprocità, senatore Amato. Soggetti giapponesi hanno già risposto, peraltro, in termini di generoso mecenatismo allo sviluppo di conoscenze specifiche sull'arte italiana. ricordi l'impegnativo progetto di diagnostica dedicato al ciclo murale di Agnolo Gaddi, avviato nel 2005 e tuttora in corso, finanziato al 50 per cento dal mecenate Tetsuyo Kuroda, tramite un accordo con l'Opificio delle Pietre Dure, favorito dal professor Miyashita sulla base di una fiducia nata da scambi di docenti e consolidata nel tempo. Quanto al valore della mostra giapponese, si rileva che il dipinto viene prestato quale opera originale, prestigiosa di Leonardo in collegamento con una mostra a carattere scientifico - come ho citato all'inizio su «La mente di Leonardo», curata da Paolo Galluzzi, direttore dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze, che rappresenta una sintesi della grande mostra tenutasi negli Uffizi nel 2006. Il luogo stesso è adeguato all'importanza della tavola, che viene accolta dal Museo Nazionale di Tokyo nella sala speciale n. 5 del padiglione principale del Museo, dove a suo tempo fu esposta «Monna Lisa». Si tratta quindi di un'ospitalità il cui altissimo livello, in termini di dignità culturale dell'iniziativa, è garantito dallo stesso Museo Nazionale. Mi scuso per qualche passaggio di pignoleria ma è stato

Sottosegretario, io la ringrazio per la puntualità e il garbo che ha usato, però, vede, sono molto insoddisfatto e amareggiato perché la mia prima interrogazione risale al 20 luglio. Sa, è un'interrogazione che avevo fatto dopo avere letto una nota di un'agenzia del 19 luglio in cui il vice *premier* e ministro per i beni culturali Francesco Rutelli rivelava di avere parlato personalmente con il sovrintendente responsabile per autorizzare il trasferimento del grande quadro finora mai uscito dagli Uffizi. Il professor Paolucci, sovrintendente allora in carica, smentì. È tutta una storia di smentite. inutile ricordarle che il direttore degli Uffizi è stato contrario fino alla fine; né lui né il sovrintendente del polo museale erano stati informati di questa decisione di trasferire l'«Annunciazione». Lei mi ha risposto qui, ma la mia amarezza è data dal fatto che la sua risposta mi giunge quando l'«Annunciazione» è già a Tokio. Allora, dopo un'interrogazione a luglio, una a settembre, una i primi di marzo, il Ministero dei beni culturali mi risponde quando l'«Annunciazione» è già a Tokio. Ringrazio. però, mentre lei è venuta qui a rispondermi, il ministro Rutelli, ai margini di un convegno a Loreto criticò una mia iniziativa, una dimostrazione plateale contro questo trasferimento, ma il ministro Rutelli ieri in televisione ha parlato dell'«Annunciazione». La ringrazio di essere venuta qui a darmi delle risposte ma le cose che lei mi ha detto in gran parte le ha dette Rutelli ieri durante la trasmissione del TG 3 «Primo Piano», condotta da Maurizio Mannoni, andata in onda alle ore 23. Vede, anche qui il ministro Rutelli sostiene che questo quadro era stato richiesto dalla Casa reale giapponese. Io farò un'interrogazione al Ministro degli esteri per sapere se ciò corrisponde al vero; possibile che ci sono sempre misteri e confusione intorno a questa vicenda?

Rutelli risponde che questo non ritiene sia il caso, dato che i tecnici hanno reputato che l'«Annunciazione» potesse sostenere il viaggio. Il problema non è lo stato di conservazione: a decidere la imprestabilità di certe opere è

non possono comunque uscire dal territorio della Repubblica italiana i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo (pinacoteca, galleria, eccetera). Ecco, l'«Annunciazione» rientra in questa fattispecie perché c'è un'apposita sezione alla Galleria degli Uffizi dedicata a Leonardo dove sono esposti l'opera «Annunciazione» e altri due quadri di Leonardo. Se si toglie l'«Annunciazione», il visitatore che va lì - dopo avere pagato regolare biglietto - non capisce nulla. Per non parlare del danno che si fa ai musei, i quali non credo possano essere ridotti ad un deposito di beni a disposizione di un Ministro che li voglia inviare a destra e a sinistra. Ad ogni modo, non è il senatore Amato che pone il problema del prestito: è la è la legge. Tanto più che la commissione che lo stesso Ministro ha istituito per l'elaborazione di linee guida per il rilascio delle autorizzazioni al prestito delle opere d'arte sostiene che occorre stilare una lista delle opere che non possono essere prestate. Il direttore degli Uffizi, da questo punto di vista, conduce da anni una battaglia, sostenendo che ci sono opere, come il «Tondo Doni» o come la stessa «Annunciazione», che assolutamente non dobbiamo prestare.

che è stato fatto il massimo per garantire condizioni di sicurezza. Lo stesso Rutelli ieri, in trasmissione televisiva, diceva che la tecnica odierna consente di rendere minimi i rischi;

nel 1939, a Milano. Nel 1940 viene trasportata alla villa di Poggio a Caiano, vicino Firenze, e poi a Camaldoli, per proteggerla, perché siamo già in guerra. Finita la guerra, il 17 giugno del 1945 torna agli Uffizi, dove è sempre rimasta. E da dove nessuno si sarebbe sognato di mandarla nel contesto nel contesto di un'esposizione merceologica. I rischi ci sono sempre; ma perché far correre dei rischi al nostro patrimonio artistico? A fronte di che? La cosa che più mi ha scandalizzato, delle recenti dichiarazioni del ministro Rutelli, è che l'invio dell'«Annunciazione», così ben protetta da teche e da strumenti, consentirà consentirà un esperimento scientifico. Noi misuriamo la possibilità di garantire la sicurezza di un'opera unica al mondo mandando l'«Annunciazione»! L'«Annunciazione» diventa oggetto di una sperimentazione scientifica sulle misure di sicurezza di un'opera d'arte! Stiamo scherzando o si parla seriamente? parla seriamente? Se si parla seriamente, allora propongo di usare, se vogliamo fare sperimentazioni, altre opere decisamente minori. Non credo che questa sia una vicenda di cui il Governo abbia molto da vantarsi, francamente. francamente. È comunque una vicenda che ha evidenziato la necessità di una *dark* *list* di opere che non possono essere prestate e che non si debbono muovere dal nostro territorio.

di accettare la valutazione vincolante dei tecnici e degli esperti, perché tanti tecnici ed esperti hanno sconsigliato questo invio.

è una grandissima tecnica, un'esperta, a lei e al direttore degli Uffizi vanno tutta la mia ammirazione per la loro competenza scientifica e per l'amore che hanno per le opere che cercano di proteggere. Anche Anche il Ministro per i beni culturali dovrebbe avere forse un po' più di amore per esse. Se mi si consente un'ultima riflessione di carattere politico‑istituzionale, questa vicenda secondo me evidenzia anche la difficoltà di far convivere nella stessa figura istituzionale il ruolo di promozione del turismo e di tutela dei beni culturali.

alla luce di questa vicenda, però, mi sono ricreduto, forse è veramente bene separare le cose. Rutelli promotore del turismo italiano fa bene a fare quello che ha fatto, perché per il nostro turismo e per i nostri prodotti, dall'olio al vino, alla moda, alla pasta (ci sono anche i produttori di pasta), è importante, se c'è l'«Annunciazione» è meglio; il Rutelli ministro per i beni culturali, che deve tutelare e garantire il nostro patrimonio, no, non la doveva mandare. Quindi, è un caso in cui le due funzioni confliggono, drammaticamente. Debbo dire

va tutto bene, però non abbiamo niente di concreto. Se faccio uno scambio, mando e ho, e quello che ho di ritorno è un qualcosa di molto concreto. Se sono soltanto cose generiche, a mio avviso abbiamo fatto un'operazione funzionale a certi interessi commerciali,

Non credo che sia stata la conclusione di una bella storia: una storia piena di silenzi, di ambiguità, di dinieghi, di persone chiama te in causa che poi hanno detto che non c'entravano nulla, una storia che vorrei un giorno scrivere. che vorrei un giorno scrivere. Spero davvero che una vicenda del genere non abbia più a ripresentarsi. In ogni caso la ringrazio, onorevole Sottosegretario: almeno lei, a differenza del Ministro, è venuta a spiegare il senso dell'operazione qui in Senato. Il Ministro, tre volte interpellato dal sottoscritto, lo ha spiegato alla televisione, lo ha spiegato fuori, però qui in Senato non è mai venuto. Lei ha dimostrato di avere un grande senso delle istituzioni e di questo la ringrazio.

la procedura cui fa riferimento l'interrogazione del senatore Eufemi si è conclusa l'8 novembre corrente con la destinazione dei viceprefetti neopromossi alle rispettive nuove sedi di servizio, individuate fra quelle gravemente carenti di dirigenti. Preciso che tali sedi erano state individuate dall'amministrazione già il 12 luglio 2005, ben prima cioè delle operazioni di scrutinio, svoltesi il 25 ottobre e 31 gennaio successivi, ed erano state portate a conoscenza dei funzionari interessati a concorrere alla promozione. I criteri adottati per l'assegnazione mirano ad una più razionale distribuzione delle risorse sul territorio finalizzata ad una migliore funzionalità degli uffici periferici, in modo da corrispondere alle accresciute esigenze operative delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e da valorizzare la loro missione quale luogo dì sintesi e di raccordo fra le amministrazioni periferiche dello Stato e fra queste ed il sistema delle autonomie. In questo quadro, con la direttiva del 19 giugno il Ministro, nell'esercizio della propria funzione di direzione politica, ha voluto indicare un criterio generale all'interno delle linee guida cui l'amministrazione dovrà conformarsi per il futuro, ma, lo sottolineo, senza entrare in alcun modo nel merito degli atti concreti di gestione. Si tratta di un indirizzo coerente con lo spirito del decreto legislativo n. 139 del 2000 di riforma della carriera prefettizia che, per sottolineare la proiezione territoriale, già prevede necessariamente per i vincitori di concorso, all'atto dell'immissione in ruolo, l'assegnazione agli uffici decentrati. Segnando una svolta rispetto al passato, esso riguarderà, con la dovuta gradualità, tutti i funzionari prefettizi e le relative future assegnazioni, allo scopo di orientare una nuova politica del personale in grado di guidare ed accompagnare l'azione dell'amministrazione nel processo in atto di trasformazione ed evoluzione delle prefetture; processo che, come noto, trae origine dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dalle successive modifiche sull'organizzazione di Governo, dal citato decreto di riforma della carriera prefettizia, che ho ricordato prima, nonché dai conseguenti provvedimenti di attuazione e modifica che hanno profondamente inciso sugli assetti e sui modelli organizzativi degli uffici di rappresentanza del Governo sul territorio. Quanto alle norme ed alle procedure specificamente applicate, si precisa che la destinazione dei viceprefetti, al termine del corso di formazione, è avvenuta in applicazione dell'articolo 12 del già richiamato decreto legislativo n. 139 del 2000, che disciplina il conferimento degli incarichi ai funzionari prefettizi. Tale disposizione regola, in via di principio, l'attribuzione degli incarichi di funzione indistintamente a tutti i funzionari prefettizi nell'intero percorso di carriera, da viceprefetto aggiunto a prefetto; essa, pertanto, non poteva non essere applicata ai viceprefetti, una volta conseguita la qualifica all'esito del corso di formazione. Ciò non toglie, ovviamente, che nei confronti dei neo-viceprefetti trovino applicazione anche le norme relative alle procedure di mobilità, così come regolate dal decreto ministeriale del 3 dicembre 2003. Nello scorso mese di agosto alcuni di essi hanno pertanto legittimamente ritenuto di avvalersi della procedura di mobilità straordinaria richiamata nell'interrogazione, esperita in applicazione dell'accordo sindacale sottoscritto il 10 luglio 2006. Tale accordo individua le sedi con grave carenza di organico da inserire nella mobilità, stabilendo un vincolo di permanenza di due anni nella nuova sede e la corresponsione ai dirigenti così trasferiti di un'indennità forfettaria pari a 1.000 euro lordi mensili. Alla scadenza del biennio, i predetti funzionari matureranno un diritto di precedenza a rientrare nella sede di provenienza o di preferenza per l'assegnazione ad una sede diversa. Tale procedura si è conclusa nel mese di settembre con l'assegnazione di 12 neo-viceprefetti ad altrettante sedi carenti; gli altri neo-promossi che non hanno ritenuto di avvalersi delle opportunità della mobilità straordinaria sono stati, invece, chiamati a scegliere, secondo l'ordine di graduatoria, la rispettiva sede d'assegnazione fra quelle gravemente carenti precedentemente individuate. detto, si è inteso realizzare l'obiettivo, di cui gli stessi funzionari erano già da tempo avvertiti, di una più razionale allocazione delle risorse in funzione di una maggiore funzionalità ed operatività degli uffici periferici; il tutto nel rispetto delle regole vigenti, nella massima trasparenza e non senza aver adottato, attraverso lo strumento della mobilità straordinaria, un sistema di offerta di garanzie, di incentivi e di compensazioni in grado di contemperare le esigenze dell'amministrazione con quelle del personale interessato. Per completezza d'informazione aggiungo infine che avverso i provvedimenti di assegnazione di cui si è detto è stato proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale in le istanze di sospensiva del provvedimento impugnato sono state rigettate in dieci casi ed accolte in tre (due dal TAR della Sicilia e uno dal TAR dell'Emilia-Romagna, quest'ultima decisione già impugnata dall'amministrazione), mentre per gli altri quattro ricorsi promossi avanti al TAR del Lazio la causa è stata avviata direttamente alla decisione di merito, non ancora intervenuta. Alcune delle ordinanze che hanno respinto le istanze di sospensiva sono state impugnate dagli interessati. In un solo caso il Consiglio di Stato ha ordinato la concessione della sospensiva, mentre altri cinque appelli proposti dalla parte privata sono stati respinti, a conferma della correttezza e della legittimità dell'operato dell'amministrazione. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Pajno per la risposta che ci ha fornito, anche se non posso ritenermi soddisfatto, per le ragioni che esporrò. Intanto, vede, onorevole Sottosegretario, l'interrogazione era del settembre scorso: abbiamo dovuto attendere oltre sei - quasi sette - mesi per avere una risposta che, semmai, presenta anche il pregio di qualche elemento ulteriore di informativa.

Ma il criterio legislativo va rispettato nella sua interezza e nella sua sostanza, perché la mobilità per prefetti e viceprefetti - avendo lei richiamato l'articolo 12

Il trasferimento per i 65 neoviceprefetti del periodo 2003‑2005 si è verificato d'ufficio, senza alcun incentivo economico, a totale discapito proprio della volontarietà - questo principio che richiamavo - e senza alcuna indicazione circa un eventuale ipotetico rientro o relativamente alle sue modalità. In particolare, tale procedura ha penalizzato 25 viceprefetti ubicati a Roma, mentre al Viminale vi erano posti liberi, sostanzialmente congelati.

quale principio generale, deve, evidentemente e uniformemente, coinvolgere tutte le categorie che rientrano nella normativa generale, indistintamente ed in modo equo. D'altra parte, rispetto a questo procedimento autoritativo, sono successivamente intervenute le circolari del 12 luglio 2005 e del 9 febbraio 2006, bandite con una procedura straordinaria, incentivate economicamente e di durata limitata. palesi, dunque, la difformità dei criteri adottati che si registra, l'estemporaneità delle decisioni assunte e la contrarietà delle stesse nei confronti della normativa in vigore.

invece, risulta estremamente attuale. Questa linea dovrebbe determinare i connotati fondamentali rispetto al prefetto, quale figura di garanzia, e trovare una linea univoca nell'aderenza ai princìpi legislativi per le decisioni future: dobbiamo favorire questa nuova fase, ripartendo proprio dal *vulnus*. Lei ha richiamato, in precedenza, un'attenzione particolare rispetto agli incentivi:

Voglio aggiungere che in gennaio vi è stato anche un incontro tra il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'economia e i sindacati per affrontare il problema della riorganizzazione del trasferimento di funzioni a livelli istituzionali. È facile osservare che nel caso che abbiamo richiamato la mobilità è stata attuata senza accordo con i sindacati, senza quella concertazione che avrebbe dovuto essere richiesta, senza incentivi e per sedi anche lontanissime. quindi, il beneficio previsto dalla legge n. 100 del 1987, peraltro insufficiente a coprire le spese reali di alloggio, secondo le indicazioni delle sedi e secondo quanto promesso dall'amministrazione, potrebbe non essere corrisposto affatto o solo con mesi di ritardo. Credo quindi, signor Sottosegretario, che vi siano moltissime incongruenze anche nella risposta che ci è stata fornita.

per venire incontro alle loro reali esigenze. Per queste ragioni, mi ritengo insoddisfatto, auspicando che per via amministrativa queste mie indicazioni possano essere recepite.

Signor Presidente, rispondo adesso all'interrogazione del senatore Di Bartolomeo sulla paventata chiusura della Scuola allievi agenti di Campobasso. Com'è noto, a seguito delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 431, della legge n. 296 del 2006 (cioè la legge finanziaria 2007), il Ministero dell'interno sta attuando un ampio piano di riassetto del «Sistema Scuole» della Polizia di Stato, sulla base di una rivalutazione complessiva del fabbisogno di formazione ed alla luce della riforma della leva obbligatoria e della figura del «poliziotto ausiliario» ad esso collegata. Ricordo che il sistema degli istituti di formazione della Polizia di Stato comprende tredici scuole per allievi agenti. La ricettività complessiva di queste scuole è di oltre 4.700 posti, ma nel prossimo quinquennio l'assunzione di nuovi dipendenti non dovrebbe superare la media di 1000 unità l'anno. Si tratta di un divario davvero consistente che, sotto il profilo del buon andamento dell'azione amministrativa, deve essere colmato sia dal punto di vista del contenimento delle spese di gestione, sia sotto l'aspetto del reimpiego del personale di polizia ivi in servizio nei compiti di controllo del territorio e di prevenzione e di contrasto della criminalità. La finalità è quella di raggiungere le necessarie economie senza, tuttavia, incidere sull'efficienza del servizio formativo. Il risparmio complessivo in termini finanziari sarà pari a circa 12 milioni di euro annui, vale a dire il 10 per cento della spesa sostenuta nel 2005 per finanziare l'intero sistema delle scuole di polizia. Verranno così conseguite le economie richieste dalla legge finanziaria per il 2007 (appunto all'articolo 1, comma 434). Alla definizione del predetto piano di riassetto si è giunti anche sulla base di una serie di incontri con le organizzazioni sindacali, alle quali, in un clima di proficuo confronto dialettico, sono state fornite precise garanzie circa la ricollocazione del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno, sia dal punto di vista logistico che sotto il profilo della valorizzazione delle professionalità. Nella scelta delle scuole da dismettere vengono prese in considerazione le dimensioni e le caratteristiche strutturali degli stabili, così come la possibilità di una loro diversa utilizzazione, ferma restando la necessità di garantire una equilibrata distribuzione territoriale degli istituti. Detto progetto di riorganizzazione dell'apparato degli istituti di istruzione della Polizia di Stato verrà realizzato in due fasi distinte. La «fase uno», la prima fase, che costituisce il primo momento di questa generale operazione di riordino del sistema, ha come obiettivo la dismissione e la contestuale riconversione di quattro scuole allievi agenti, per un totale di circa 900 posti letto. La «fase due» prevede un passaggio successivo e cioè la dismissione di ulteriori tre scuole allievi agenti da individuare in una rosa di nove istituti, per un totale di 1.300 posti letto. Per quanto riguarda, in particolare, la Scuola di Campobasso, comunico che essa è inserita nella «fase due» ed è pertanto uno dei nove istituti nel novero dei quali saranno scelte le strutture da chiudere. Preciso però che al momento per tale istituto nessuna decisione definitiva è stata ancora assunta. In astratto, l'ipotesi di dismissione della struttura potrebbe tuttavia ritenersi in qualche modo giustificata dalle ridotte dimensioni del complesso (236 posti letto) e dalla possibilità di una proficua riconversione in favore della Questura e del compartimento locale della Polizia postale e delle comunicazioni, uffici che presentano una inadeguata situazione logistica. Ritengo infine opportuno precisare che l'eventuale soppressione dell'istituto, che - ripeto - non è ancora stata deliberata, non penalizzerebbe l'area geografica di riferimento, in quanto rimarrebbe in funzione la vicina Scuola allievi agenti di Caserta,

tra quelle di proprietà dello Stato. A me risulta - non so se le indicazioni sono sbagliate - che addirittura il Ministero dell'interno usi locali in fitto da privati per tenere le scuole di Polizia di Stato. Allora, se è vero che dobbiamo andare verso una ristrutturazione e un'economia, non mi pare giusto togliere una scuola, peraltro nuova, costruita nel 1996 dallo Stato, e attrezzata in tutti

e antisismica. Lo Stato ha speso soldi per formare il personale di quella Scuola perché, mentre faceva formazione, non faceva servizi. Le posso assicurare che i 59 agenti

verrebbero chiuse unitamente alla Scuola. Il problema del personale di polizia del compartimento delle poste, poi, non è vero:

partecipato al «pellegrinaggio» presso il Ministero dell'interno insieme a qualche deputato, al Sindaco di Campobasso e al Presidente della Provincia di Campobasso. Era questa la sede dove il senatore Massa doveva

per avere visibilità nella mia Regione (sono 35 anni che faccio politica, ho rivestito tutte le cariche che in Regione vi sono, da Presidente della Giunta in poi): sono qui per chiederle proprio, come cittadino e molisano, di non toccare quella struttura; è un gioiello

più il danaro per mantenere quella scuola. Badi bene, signor Sottosegretario, che stiamo parlando di 100.000 euro l'anno (tanto è il costo di gestione

dell'Unione Europea un progetto per una Scuola di criminologia, che potrebbe trovare ubicazione e logistica in quell'edificio. La Regione e la Provincia insieme